nella seduta antimeridiana di oggi ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e sono stati votati gli stralci agli articoli 5 e 6. Ricordo Ricordo che il voto finale dell'articolo 2 è stato accantonato. Sono stati altresì accantonati l'emendamento 3.800 del Governo, per l'esame da parte della 5a Commissione, e il voto finale dell'articolo 3.

Grazie,

Non ci siamo proprio. Arriveremo a una o due votazioni dove, se non siete seduti e non c'è silenzio, non farò votare.

Presidente, Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 4.101, esplicativo di una posizione che, per ipocrisia legislativa o per timore di chi non vuole che gli avvocati abbiano un componente di diritto nel consiglio direttivo della Cassazione, non verrà appoggiato da tanti. Vorrei però rivolgermi agli avvocati agli avvocati presenti nel centro-sinistra: con quale faccia andrete poi a dire al vostro Consiglio dell'ordine che non volete il presidente del Consiglio nazionale forense componente di diritto del comitato direttivo della Cassazione? Qui non si difendono posizioni particolari, si dà un giusto riconoscimento al vertice della vostra categoria.

nel Consiglio direttivo della Cassazione. Poi non venite a raccontare alla vostra categoria che si votava solo per ragioni di coerenza di coalizione; qui è un'altra storia. Non c'entra nessuna coerenza di coalizione, qui non c'è né destra, né sinistra, c'è soltanto una logica giustamente premiale di rappresentanza a favore di una categoria. Presidente, immediatamente dopo vi è il mio emendamento 4.102, di fatto identico a quello che stiamo per votare. Vorrei evitarne la preclusione e annuncio al collega Centaro che anche noi voteremo a favore del suo emendamento

strutturalmente questa legge ha due grandi nemici: gli italiani e gli avvocati. Gli italiani li abbiamo già sistemati con gli altri tre articoli; gli avvocati vengono sistemati come sudditi con l'articolo 4. Quindi, voteranno contro sapendo che questa legge è contro gli italiani e contro gli avvocati.

consentitemi, egregi colleghi, di svolgere alcune considerazioni. Piero Fassino, il segretario politico dei DS, in alcune interviste televisive trasmesse ieri sera e questa mattina, ha accusato di irresponsabilità politica chi, con proposte emendative, ha creato o crea fibrillazioni al Governo. Mi dispiace molto questa sua valutazione perché ho grande, grandissima stima di lui. Devo però ritenere che parla senza conoscere bene i fatti, forse perché i nuovi sergenti della politica che costituiscono la classe dirigente parlamentare probabilmente lo disinformano, quanto sono ancora così autoreferenziali e pregni di centralismo democratico da non riuscire a considerare con il dovuto rispetto i valori repubblicani di una libera ed autentica democrazia parlamentare partecipata. Quello stesso centralismo democratico che ha indotto, ad esempio, signor Presidente, il vertice del Gruppo dell'Ulivo a dichiarare il voto contrario sul mio emendamento senza convocare preventivamente alcuna assemblea di Gruppo. Ma tant'è. Sul merito dell'emendamento ho poco da dire, giacché la proposta che faceva parte del testo finale del Comitato ristretto, votato favorevolmente - sottolineo, votato favorevolmente - da tutta la maggioranza, era stata discussa ed approvata in Commissione. Per fortuna, la rassegna stampa quotidiana di oggi ed i resoconti parlamentari dei giorni scorsi danno conto di come tale soluzione all'epoca fosse condivisa in Commissione, fra gli altri, ad esempio, da tre valenti magistrati parlamentari, i colleghi D'Ambrosio, Casson e Di Lello. E questa valutazione mi serve per dissolvere ogni sospetto di arcaico ostracismo preconcetto della magistratura illuminata nei confronti dell'avvocatura. Ed allora forse dovremmo tutti chiederci perché i Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati prima vengono considerati da tutti - e dico da tutti, opposizione compresa - quali legittimi componenti di diritto dei Consigli giudiziari e poi, invece, vengono di fatto eliminati. Se le legittime rappresentanze parlamentari di tutti i Gruppi, alla fine di un percorso, Presidente, che è stato argomentato e condiviso nel merito, riconoscono la legittimità di tale scelta, perché perché il Parlamento sovrano deve subire le pressioni e i ricatti di segno opposto che vengono dall'esterno? Questa domanda aleggia ed aleggerà in quest'Aula. Presidente, quando iniziammo, nel mese di settembre dell'anno scorso, l'esame del primo provvedimento del Governo sull'ordinamento giudiziario - ricordo in particolare che si stava per decidere sulla sospensione di uno dei decreti legislativi del senatore Castelli, che regolamentava l'organizzazione delle procure - io ebbi il coraggio di affermare in quest'Aula che avrei votato un emendamento dell'opposizione (mi pare di ricordare fosse un emendamento del collega Caruso), che rendeva invece effettiva quella riforma. mettendomi nei panni del cittadino comune, mi sarei sentito più tutelato dal nuovo modello di organizzazione piramidale delle procure che, facendo capo direttamente al procuratore, rendeva condivise le indagini, evitava la spettacolarizzazione spettacolarizzazione delle inchieste e sottoponeva le richieste di misure cautelari ad un più rigido controllo. Ci fu un momento di sconforto, come forse quello che vive l'Assemblea in questo momento; poi,

che ci portò ad approvare le modifiche di due decreti legislativi su tre, sospendendo l'efficacia soltanto di quel decreto legislativo che è oggi all'esame del Senato. In quel modo, signor Presidente, recepimmo ed applicammo quel concetto di condivisione che il Capo dello Stato ci ha chiesto sempre di privilegiare per l'approvazione di provvedimenti complessi e delicati, quale è quello sulla giustizia, che non possono risentire di un clima ostile di contrapposizione preconcetta. Allora, mi pare di ricordare, il ministro Mastella fu il primo a condividere questi principi. Il confronto, onorevoli colleghi, la condivisione, la partecipazione democratica, il rispetto delle libere e consapevoli decisioni delle Commissioni e dell'Aula sono valori che dovrebbero appartenere al bagaglio culturale di tutti i parlamentari; l'Assemblea è libera e sovrana e io sono pronto ad accettarne il responso, senza retropensieri, senza furbizie e senza mercanteggiamenti. Se il mio emendamento dovesse essere bocciato, ne sarei dispiaciuto perché sarebbe un'ingiustizia enorme consumata in danno di tutta l'avvocatura, ma non ne farei un dramma. Con la stessa logica, se il mio emendamento dovesse essere invece approvato, chiedo a lei, ministro Mastella, di prendere atto che quello sarebbe un voto a favore della presenza degli avvocati e non contro il Governo, che non può

purtroppo viene strumentalizzata per assurde lotte tribali. Mi piace concludere, Presidente, precisando per i tanti apprendisti stregoni che mi ascoltano, e che hanno immaginato dietro i miei comportamenti chissà quali sordide manovre, che, insistendo nel voto, non voglio difendere la mia proposta per un eccesso di edonismo politico, ma voglio salvaguardare l'essenza profonda delle istituzioni democratiche da noi rappresentate, che devono rimanere consapevoli del loro ruolo

discussioni di questa natura vennero fatte addirittura su voti di fiducia; caddero Governi. Se guardiamo poi, nel dipanarsi del *fil rouge* della storia repubblicana, di fatto non accadde nulla di gravissimo, ma semplicemente vennero esercitate le prerogative costituzionali e democratiche del Paese, al di là poi, magari, dei drammi personali dei singoli. Quindi, oggi siamo in una situazione interessante, ma non di particolare gravità. Qual è la peculiarità di questa situazione, signor Presidente?

il modo di superare questo momento di difficoltà della maggioranza e del Governo fosse quello dei metodi tradizionali, con le riunioni, con le convocazioni, con le proposte di mediazione, con la ricerca di un testo condiviso: questo fa parte della fisiologia del gioco democratico. Ebbene, che cosa accade oggi, in quest'Aula? Torniamo nella patologia. Come pensa, infatti, l'Ulivo di superare questa sua *impasse* interna? Chiama le forze di coloro i quali non sono mai stati eletti da nessuno. Questo è sbagliato, signor Presidente. Per favore, non venite a dirci che hanno diritto di votare, lo sappiamo, ma qui ci sono alcuni sconfitti, signor Presidente. Il primo sconfitto è il popolo italiano. Certo, il popolo italiano, perché voi non siete qui perché siete bravi, belli e intelligenti (nemmeno noi), ma perché vi ha mandato il popolo e state qua finché siete in grado di starci, sulla base del voto popolare. Se non ci riuscite, è bene tornare di fronte al popolo e votare. No, voi invece chiamate le truppe di rinforzo. Ora, io distinguo perfettamente il ruolo del senatore Andreotti da quello degli altri senatori a vita, perché il senatore Andreotti è sempre presente, svolge il suo ruolo di senatore a vita in maniera completamente autonoma ed è sempre qua. Credo che lo spettacolo costituzionalmente, istituzionalmente e formalmente corretto di senatori a vita che vengono qui semplicemente perché la maggioranza non è in grado di risolvere i propri problemi,

per voi che scendete un altro gradino nella vostra dignità, perché non siete capaci di comporre le contraddizioni al vostro interno e allora chiamate delle persone terze, che vengono a darvi, dire, un vantaggio temporaneo, assolutamente temporaneo. Ma le vostre contraddizioni resteranno. Infine, mi rivolgo a lei, dottoressa Montalcini. Lei è stata nominata in forza dell'articolo 59 della Costituzione. Lei ha avuto altissimi meriti in campo scientifico, artistico, letterario e così ha illustrato la Patria. È sicura che in questo momento, venendo a votare a comando, lei illustra la Patria? Le faccio una domanda accorata: ma perché lei, che era una persona ammirata da tutto il popolo italiano,

Presidente, leggendo e rileggendo l'emendamento scritto dal senatore Manzione, mi chiedevo dove avessi già udito una proposta del genere. Per fortuna c'è qui il senatore Buccico, che contrasta efficacemente il mio Alzheimer incipiente. Ebbene, questa proposta, che

di modifica dell'assetto dell'ordinamento giudiziario redatto dalla formazione di Magistratura democratica, la corrente di sinistra (non proprio di estrema sinistra, ma insomma di sinistra consolidata), la corrente comunista dell'Associazione

l'Associazione nazionale magistrati sia poi così invasiva nei confronti del Parlamento se è vero, come è vero, che la maggioranza di centro-sinistra oggi si appresta, salvo colpi di scena, a votare compattamente contro l'emendamento del senatore Manzione. No, vuol dire semplicemente che l'accorta politica, la scaltra politica dei magistrati di Magistratura democratica in un certo momento ha loro consigliato di inserire una proposta che fosse in qualche maniera evocativa di qualcosa di gradito ai magistrati. Insomma, è per dire che, anche sulle cose che possono avere un senso logico, un contenuto di messaggio forte nei confronti di coloro che della giustizia si servono, questi signori si pongono pur sempre, e per sempre, in maniera assolutamente strumentale, in maniera semplicemente scaltra. E non voglio assolutamente dire, senatore Manzione, che la sua proposta è figlia di una identica, di una analoga, di una simile logica, perché sono testimone di quello che si è detto, di quello che si è discusso, degli argomenti che sono stati posti nel lavoro della Commissione giustizia del Senato e so che la costruzione che il suo emendamento, senatore Manzione, evoca era il frutto di condivisione, era il frutto di ragionata condivisione. Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento per due ragioni. Voterà a favore di questo emendamento perché è una soluzione legislativa che genera armonia nell'ampio perimetro del sistema che rende giustizia ai cittadini. Voterà a favore di questa proposta perché è la proposta di un uomo libero, che ha saputo dimostrarsi libero.

chi sono gli uomini liberi, chi sono i sudditi perché sudditi, o sudditi per convenienza.

Presidente, ci accingiamo a votare un emendamento che faceva parte di quel pacchetto di proposte approvate dalla Commissione. Un emendamento che prima era condiviso dalla maggioranza, credo dal Governo, e che oggi viene contrastato da una maggioranza che, essendo in difficoltà nei suoi numeri, chiede il soccorso rosso dell'armata di riserva dei senatori a vita, arrivati poc'anzi in quest'Aula anche se non hanno mai seguito alcunché di questo dibattito né in Commissione, né in Aula. e LNP)*. Ricordo il comunicato del Capo dello Stato durante le consultazioni relative alla crisi apertasi a seguito delle dimissioni dell'attuale Presidente del Consiglio: ebbe a rimandare il Presidente del Consiglio alle Camere perché verificasse se quel Governo avesse o meno una maggioranza politica in Parlamento.

Cosa succede oggi, signor Presidente? Alla luce degli eventi di ieri e del fatto che il ministro Mastella ha preso atto, di quell'onestà intellettuale che gli riconosciamo, che non aveva più una maggioranza tale da indurlo a rimettersi all'Aula su tutti gli emendamenti su cui esprimeva il parere, per evitare di essere «bruciato», egli ha riconosciuto di non avere la certezza di una maggioranza in Aula.

Ieri si è realizzato uno strappo: la maggioranza politica in Aula non c'era, abbiamo assistito a dichiarazioni, minacce, controminacce, lettere paventate di dimissioni di un Ministro nei confronti del Presidente del Consiglio e visite in Senato dell'onorevole Fassino per occuparsi di questo tema. Insomma, una crisi politica vera, non soltanto parlamentare. Allora oggi cosa si consuma, signor Presidente? Per evitare che si possa realizzare in quest'Aula anche una crisi parlamentare - perché la crisi politica già c'è - si chiede il soccorso numerico - squisitamente numerico a parlamentari di quest'Aula che, non avendo una legittimazione popolare, sono in grado di sovvertire una crisi politico-parlamentare che ieri si è aperta. Allora, vedete - colleghi - mi chiedo e chiedo perché questi illustri senatori a vita, un ex Presidente della Repubblica, una scienziata di chiara fama, si prestino a sostenere un Governo nel quale non sono stati eletti per il cui sostegno non hanno avuto il consenso dei cittadini; un Governo che gli stessi cittadini italiani ormai hanno chiaramente manifestato, in occasione di tante tornate elettorali, di voler mandare a casa per il semplice motivo che li ha delusi. Me lo chiedo e ce lo chiediamo: signor Presidente, registriamo un'ulteriore crisi della politica del Paese, di un sistema sostenuto soltanto su voti raccattati all'ultimo minuto, come allarme rosso, per sostenere una realtà istituzionale, quella dell'Esecutivo del Presidente del Consiglio, che ormai ha fallito il proprio progetto. Basta leggere, colleghi, i giornali di oggi, di centro‑destra e i grandissimi e numerosissimi giornali di centro‑sinistra: uno per tutti, quel famoso giornale - il più importante d'Italia - che in campagna elettorale con un editoriale aveva invitato a votare Prodi. Leggetelo oggi e vedete cosa dice di voi! Ebbene verificheremo tra poco quello che succederà. Alla luce di quello che succederà, trarremo le nostre conseguenze, perché, signor Presidente, non le nascondo che cominciamo a essere stanchi di questa situazione. Continueremo ugualmente a condurre la nostra battaglia, perché sappiamo che ormai manca poco, molto poco, alla caduta di questo Governo, un Governo che cadrà in quest'Aula come è caduto la prima volta.

il Gruppo dell'UDC si muove lungo la linea indicata dal collega Manzione al quale intendiamo attribuire un grande merito, l'aver pronunciato stasera in Aula Aula parole di estrema chiarezza: non è in gioco il rapporto maggioranza-opposizione, non è in gioco il rapporto di coerenza della maggioranza all'interno di proprie componenti, è in gioco il problema della libertà di questo Parlamento nei confronti di soggetti esterni. Siamo particolarmente grati al collega Manzione, perché mi auguro che, all'interno dello schieramento politico del quale egli fa parte e desidera continuare fare parte,

è in gioco il significato che intendiamo attribuire ad una scelta che la Commissione giustizia aveva già ritenuto adeguatamente tale da parte della maggioranza dell'opposizione. La Commissione giustizia, in un certo senso, aveva già dimostrato che - contrariamente a quanto ho detto più volte in quest'Aula - non vi era un intendimento dei magistrati contro gli avvocati. Il collega Manzione ha ricordato il contributo decisivo

voti compatta a favore dell'emendamento, perché in questo modo dimostrerebbe che non è in gioco il rapporto tra maggioranza opposizione, ma - come ho detto e ripeto - la novità che questo Parlamento potrebbe esprimere ed è chiamato ad esprimere. Grazie, Manzione.

Signor Presidente, volevo soltanto richiamare la sua attenzione - sempre notevole - sul fatto che il Presidente dell'Assemblea non dovrebbe permettere, nei confronti dei senatori e delle senatrici a vita, parole come "voti raccattati" oppure le offese che, ancora una volta, abbiamo sentito in quest'Aula.

signori del Governo, onorevoli colleghi, non ci sfugge certamente, e non sarò io a negarlo, che fra le ragioni del voto che mi accingo ad esprimere ci sono le difficoltà politiche del Governo che sostengo, difficoltà che esistono in Senato fin dall'inizio della legislatura, per le ragioni numeriche che conosciamo e che si aggravano nel rapporto con il Paese nelle difficoltà ad affrontare i problemi che lo stesso ha di fronte. Tuttavia, rivendico, senza aver bisogno di citare Max Weber e l'etica della convinzione e l'etica della responsabilità, che tra i motivi di scelta di un parlamentare, al momento del voto, pur rispettando la diversa decisione del collega Manzione, c'è anche quello di valutare gli effetti che il suo voto può produrre sulla sopravvivenza o meno del Governo che sostiene. Tanto più quando ci troviamo di fronte ad una norma che (vorrei spiegarlo ai colleghi, perché conviene richiamare l'attenzione sui contenuti) è certamente diversa da quella contenuta nel testo originario forse soddisfa anche meno, non voglio sottacerlo, un'esigenza alla quale personalmente ho creduto da tempo e alla quale un tempo credevano anche i settori più avanzati della magistratura italiana (ma sull'interlocuzione con quest'ultima mi pronuncerò al momento della dichiarazione di voto): la presenza cioè dei laici nei consigli giudiziari. E tuttavia non si può dire che il testo che abbiamo trovato in Commissione non venisse incontro al problema, che pure esiste, di assicurare agli avvocati, che garantiscono nel Paese

prepotenti, prevaricatori, inerti, corrivi o disonesti, la loro voce potesse pesare. Nel nuovo testo che abbiamo introdotto, e che io difenderò esprimendo il voto contrario alla proposta del senatore Manzione, è vero che non è stata più prevista la presenza degli avvocati laici nei consigli giudiziari; è vero però che si è modificato un altro punto molto rilevante della legge, che i colleghi troveranno nella lettera *f**)* del comma Che cosa abbiamo previsto per controbilanciare il venir meno della presenza degli avvocati nei consigli giudiziari? Mentre il testo originario prevedeva, appunto perché c'erano gli avvocati nei consigli giudiziari, che i capi degli uffici, nel fare rapporto al Consiglio superiore della magistratura, potessero o meno tener conto delle segnalazioni provenienti da cittadini o da avvocati, noi abbiamo dato un ruolo formale e autonomo alle segnalazioni formulate dal consiglio dell'ordine degli avvocati, «sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica». Per la prima volta, quindi, nell'ordinamento giudiziario italiano viene introdotto il principio per il quale il rapporto del consiglio dell'ordine in quanto tale - quindi, non del singolo avvocato su un magistrato, che segnali specificamente questi elementi ai quali ho fatto riferimento, assume un ruolo e una funzione autonoma rispetto al rapporto del capo dell'ufficio; tant'è vero che si dice nel passaggio successivo: «Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario (...) e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura», il quale nel deliberare non potrà non tenerne conto, se non altro per il principio del diritto amministrativo per il quale, qualora il Consiglio superiore della magistratura non tenesse conto di questo parere, il provvedimento sarebbe carente per difetto di motivazioni e impugnabile davanti al tribunale amministrativo regionale. Io quindi credo i che chi vorrà esprimere, come io invito a fare, voto contrario all'emendamento Manzione, troverà nell'ordinamento giudiziario ciò che più ci interessa, cioè una norma che garantisca anche all'avvocatura, nella sua espressione formale, che è il consiglio dell'ordine, di far valere i comportamenti negativi della magistratura con un rilievo e con un'incidenza

Signor Presidente, io non mi soffermerò sul contenuto tecnico dell'emendamento, perché lo hanno fatto meglio di me

è una buona proposta, che fino a quand'è stata in bocca all'allora ministro Castelli è stata contestata con forza e per principio, forse perché veniva da quella parte, una cosa che in bocca al senatore Manzione comunque è condivisa anche da altri, ancorché votino contro. Insomma, una richiesta intelligente, condivisibile non solo da noi ma, in modo più vasto, da parte dell'Aula; pare quindi che ci sia un ordine di schieramento, un ordine partitico: non ho mai usato questa parola, ma la voglio usare per chi a partiti non appartiene, come la dottoressa Rita Levi Montalcini, come altri senatori a vita, quale Pininfarina, che non è presente, a cui volevo scrivere una lettera aperta, come sanno bene i componenti della Commissione lavoro, che con sorpresa l'altro giorno sono stati messi in minoranza dal voto

da un collega del Gruppo Misto. Ora, cosa volevo scrivere nella lettera a Pininfarina, che sicuramente è un che sicuramente è un grande uomo dell'industria italiana, un cavaliere del lavoro, che ha espresso più volte, nella fattispecie di cui parlo, degli orientamenti chiari, come per esempio il sostegno totale alla proposta poi diventata legge Biagi? ma il giorno in cui verrà qualcuno a sostituirlo e a sostenere - credo a sua insaputa - esattamente il contrario in Commissione, non staremo operando un *vulnus* proprio contro la democrazia e contro la Costituzione?

che appartengono a forze politiche non lo trovo democratico, né liberale. Pertanto, è chiaro che anch'io seguirò

Signor Presidente, nel merito dell'emendamento e sulle valutazioni per cui esprimiamo voto contrario,

soltanto su un punto politico di grande rilevanza. Vorrei rassicurare il senatore Caruso, il senatore D'Onofrio e anche il senatore Manzione sulla libertà del Parlamento sulla libertà di voto di ogni singolo e singola parlamentare. Ognuno di noi infatti esprime un giudizio politico nel merito, ma anche un giudizio politico sulle condizioni di equilibrio tra il voto su una singola norma, come questo emendamento, e il senso e il merito complessivo del provvedimento, nonché sui rapporti politici. Considero un valore politico la costruzione della mediazione, dell'accordo nel confronto esplicito, come è avvenuto intorno a questo provvedimento in tutti i suoi passaggi, e non accetto da parte di nessuno lezioni su libertà e democrazia. Vorrei ricordare al senatore D'Onofrio Kelsen, un teorico liberale che per me ha fatto scuola e sul quale insegno ai miei studenti il senso della democrazia parlamentare, ritiene parlamentare, ritiene che la mediazione è la funzione del Parlamento e che la ricerca della mediazione politica non è una vergogna, ma un valore politico. Non mi sento dunque costretta, vincolata, né condizionata. riterrò questa mediazione in qualche modo non compatibile con le mie convinzioni profonde, la metterò esplicitamente in discussione; fino a quel momento la rivendico come una scelta politica che non consento a nessuno di tradurre in mercato, in vincolo, in coercizione, in obbedienza a poteri od organi esterni a quest'Aula. altresì a rispettare davvero chi sta fra noi perché è stato designato dal Capo dello Stato e a non affermare che anche quel voto sia dato non in coscienza, ma soltanto in obbedienza,

con molta tranquillità, vorrei sfrondare subito qualsiasi forma di polemica.

Presidente. Siccome noi vogliamo rimanere in un sistema di libera democrazia partecipata, ma qui c'è il rischio che si finisca in un sistema di libera democrazia pilotata, le chiedo di far allontanare la collega Soliani

poiché ci troviamo di fronte ad un emendamento di particolare complessità, ritengo utile avvertire l'Assemblea sugli esiti procedurali derivanti dalla votazione dell'emendamento 4.106 del Nel caso di reiezione, non vi sono effetti preclusivi sugli emendamenti successivi. Nel caso di approvazione, risultano assorbiti gli emendamenti 4.107, 4.108 e 4.109,

Signor Presidente, in questi giorni, in questi giorni, i colleghi della Commissione di merito, Buccico, Valentino e, in modo particolare, il collega Caruso, hanno affrontato questo hanno affrontato questo provvedimento con grande senso di responsabilità. Da martedì, in Aula, abbiamo affrontato il provvedimento con altrettanto senso di responsabilità. Ci siamo confrontati in un dibattito civile, in alcuni momenti anche duro, ma certamente abbiamo poi rispettato il voto che l'Assemblea ha espresso. Abbiamo quasi sempre perduto, escluso in un'occasione, ma certamente abbiamo partecipato, come sempre, alla vita democratica nell'approvare un provvedimento legislativo.

È capitato a tanti di noi, su alcuni provvedimenti, di essere isolati o, comunque, minoritari all'interno anche del proprio Gruppo. È capitato anche a me. Ricoprendo il ruolo di Presidente del Gruppo, sono stato in grande imbarazzo quando si è approvato in quest'Aula l'indulto: il mio partito, i colleghi del mio

C'è un Capogruppo che, dopo una votazione importante, ha chiesto la parola. La regola che seguo è quella che un Capogruppo di tutti e due gli schieramenti parli brevemente: questa è una regola che dura da un pezzo.

è capitato anche a me quello che ora è accaduto al collega Manzione: succede quando siamo di fronte alla nostra coscienza e, non condividendo un provvedimento, sentiamo la forza di votare come la pensiamo. Non c'è nulla di eroico in tutto questo. Il collega Manzione ha svolto, come è giusto che faccia un parlamentare, il suo ruolo. Il collega D'Onofrio glielo ha riconosciuto poc'anzi. Non è nemmeno nel mio modo di agire l'essere irriguardoso nei confronti dei colleghi senatori a vita. Essi sono in quest'Aula o per volontà costituzionale o per meriti scientifici o politici, però, quello che si è consumato poc'anzi è inaccettabile...

Presidente, sarebbe veramente non poco rispettoso del sottoscritto e del Gruppo se la colpa fosse mia perché sto parlando troppo! PRESIDENTE Nessuno le dà colpa. Prego, intervento non vuole essere nemmeno irriguardoso: i colleghi senatori a vita fanno parte di quest'Aula per volontà costituzionale o per meriti scientifici, quindi, il loro voto è legittimo. Ma in Commissione su questo argomento non sono mai andati; in Aula, è da martedì mattina che discutiamo il provvedimento, non si sono mai presentati; sono arrivati ora, quando c'era un pericolo per il Governo. Questo Governo - è legittimo dirlo da parte di noi dell'opposizione - si regge, ancora una volta, per volontà dei senatori a vita, che hanno diritto di stare qui, ma non hanno

abbandona l'Aula, preso atto del fatto che in essa non c'è più una maggioranza politica, perché il voto dei senatori a vita è stato determinante. Di ciò prendano atto il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio, perché non ci stiamo più ad effettuare votazioni falsate sotto il profilo democratico! Mi scusi, Presidente, credo che chi ha trasformato l'emendamento in ordine del giorno avrebbe avuto il diritto di parlare prima degli interventi precedenti e lo chiedo rispetto ai colleghi dell'opposizione. Credo che questo emendamento sia stato caricato

che nel consiglio giudiziario, organismo di indirizzo, nulla di più, per chi vive il tribunale, abbia ragione d'essere la voce della magistratura (sono i gestori della giustizia a quel livello), così come abbiano ragione di esistere le voci dall'avvocatura. Quindi, proprio per andare al di là del significato politico (non deve cascare nessun Governo con questo ordine del giorno), si vuole dare un indirizzo all'Esecutivo che in quella sede debba esserci anche la voce degli avvocati, che vivono tutti i giorni in quel palazzo? Io credo sia Ho presentato un ordine del giorno, nulla di più, non cascherà niente con quest'ordine del giorno; ma vogliamo da quest'Aula dare un indirizzo che viene dal buon senso, al di là delle collocazioni politiche?

Quell'appello non è stato raccolto. Si è registrata in quest'Aula una drammatica rottura costituzionale, non politica. Il Gruppo UDC va via. *(Applausi dai Gruppi Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana-Partito repubblicano-Movimento popolare per l'Autonomia osserva con grande preoccupazione ciò che è avvenuto, in queste ore, nell'Aula del Senato. Vorrei cogliere l'occasione per sottolineare che i nervosi scambi di battute avvenuti stamane tra il senatore Bettini e la senatrice Bonfrisco in occasione dell'intervento del senatore sono uno spaccato che potremmo mandare a reti unificate per raccontare al Paese la straordinaria occasione perduta, che ancora una volta la classe politica registra al suo passivo, per non essere stata capace di riunificare il Paese in una riforma vera

la voce di un collega, stimabile e anche simpatico, che ha avuto la sciagura di rappresentare, però, il ricordo in quest'Aula di una stagione ancora viva e dolorante, se ha suscitato tante passioni e tante reazioni. In fondo a queste giornate così buie vi è stato un voto durante il quale un senatore della maggioranza denunzia il clima illiberale di un Parlamento pilotato, richiama un centralismo democratico che non viene rinfacciato all'Unione da nessuno del centro-destra. Il presidente Berlusconi ha partecipato al congresso del Partito democratico salutando come un fatto positivo la nascita di quel partito, che archivia la trilogia, a cui eravamo affezionati, del PCI, PDS e DS. Abbiamo appreso con dolore in questa'Aula che la nostra archiviazione è stata frettolosa perché un senatore del neonato Partito democratico oggi ci annuncia - e questo dibattito lo conferma - che un filo di centralismo democratico è vivo e vegeto ancora in quei dintorni.

Marini, possiamo richiamare il risultato: 155 favorevoli, 156 contrari, 2 astenuti; il dato numerico dice che il voto dei senatori a vita è determinante.

avendo rispolverato per il mio Gruppo la denominazione di Democrazia cristiana. Guardando ai senatori a vita, oltre al rispetto, non posso che avere anche la speranza di qualche resipiscenza, per cui che Dio ce li custodisca a lungo e votino come credono, ma sia chiaro un dato politico:

- e il Parlamento, in uno dei suoi due rami, si regge sul voto determinante dei senatori a vita. Il Capo dello Stato, che abbiamo imparato ad apprezzare e a stimare sempre di più in questo anno di mandato, ha risolto una crisi di Governo indicando alla maggioranza la condizione ineludibile della sua autosufficienza rispetto ai senatori a vita. Questa condizione è venuta meno; è la ragione per cui vogliamo denunciare in modo forte e chiaro al Paese il cambiamento politico e istituzionale che è avvenuto oggi in Senato,

semplicemente legata a quell'istinto di sopravvivenza presente in ogni essere umano. È chiaro però che ormai, dal punto di vista politico, ma soprattutto democratico, siete arrivati alla frutta. Se siete Se siete costretti a chiamare delle anziane signore affinché vengano a votare, tra l'altro sempre assistite da senatrici che non si sa se siano veramente senatrici o badanti, lo spettacolo che date al popolo italiano

cui il senatore Calderoli

a valutare per il futuro la possibilità di iniziative legislative volte a recepire il contenuto dell'emendamento 4.106».

la parola «legislative», e quindi la possibilità per il futuro di iniziative volte a recepire il contenuto dell'emendamento 4.106, lo si può accogliere come raccomandazione.

Manzione è un senatore mio amico, che io ho contribuito, anzi determinato, a portare in Parlamento, perché ne riconosco le capacità. devo anche dire che non mi sono mai interessato di questioni di giustizia, nel senso dell'apprensione che vedo crea e porta avanti, però, quando sento espressioni apodittiche,

all'allora maggioranza - "di un provvedimento, quello del senatore Castelli, che speriamo di riuscire a bloccare", e lo diceva per conto della Margherita. "È chiaro il tentativo" - proseguiva - "di svuotare il ruolo del CSM con misure che ledono il principio dell'autonomia. Pensiamo solo alle funzioni tolte al CSM e" - badate bene - "attribuite ai Consigli giudiziari dove, guarda caso, entreranno anche avvocati e rappresentanti regionali che dovranno decidere su aspetti della carriera dei magistrati. È evidente che il Governo alla maggioranza di allora - "vogliono completare il disegno di insidiare l'autonomia e l'autogoverno della magistratura, cominciato con la riduzione del numero dei componenti.

Signor Presidente, sono lieto che i toni in quest'Aula siano scesi. Credo di poter accogliere l'invito del relatore, in base al quale egli esprime parere favorevole, e il parere del Governo che si rimette all'Aula. Ricordo quando detto, senza sottolinearne nuovamente i toni, dal collega Buttiglione: il nostro è un sistema accusatorio e quindi deve esserci un procuratore che interviene per difendere la sicurezza del cittadino rispetto a determinati reati; un giudice che rappresenta chi deve bilanciare la parte ed emettere un giudizio, e, tra queste parti, c'è anche una difesa. Quindi, come linea di indirizzo, credo che la difesa debba essere rappresentata da dove si stabiliscono non le regole ma l'indirizzo di un tribunale, senza alcunché togliere a qualunque tipo di autonomia. Ringrazio il

ad una condivisione di tutti di questo principio. Lo ha ribadito tre volte nel suo intervento, lasciando intendere che tutti i Gruppi presenti in Commissione avessero condiviso quell'impostazione. L'Italia dei Valori non l'ha mai condivisa,

Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani. Anche noi voteremo contro questo ordine del giorno, perché crediamo che oggi in quest'Aula

(non sereno, come è stato detto da diversi esponenti dell'opposizione) e soprattutto per tentare di sanare i ripetuti insulti a cui sono stati sottoposti in particolare i senatori a vita. Signor Presidente, in continuità con il voto contrario espresso sull'emendamento del senatore Manzione, confermiamo il nostro voto contrario sull'ordine del giorno presentato dal senatore Calderoli.

Lo spieghi brevemente, per favore. Tanto la sua libertà non è in discussione. PALUMBO *(Ulivo)*. ...che ritenevo, in linea di principio, condivisibile l'emendamento presentato dal senatore Manzione e che tuttavia, avendo assunto la questione (come è stato anche bene illustrato dal senatore Salvi) una valenza politica di particolare rilievo,

col voto. Le leggi sono scritte. C'è solo da dire se esiste o no il diritto ad una difesa, ad avere degli avvocati che dicano la loro. Punto. «Il Senato impegna il Governo a valutare per il futuro

**Il Senato non approva.**

Il ministro Mastella sa bene che se ci recassimo in emeroteca a rivangare e rileggere i suoi discorsi e le sue affermazioni

Per quanto riguarda la coerenza, vorrei ricordare che Magistratura democratica negli anni Settanta era collocata su posizioni opposte quelle che attualmente occupa: allora era una corrente della magistratura libertaria, una corrente che voleva portare dentro

quella figura del decisore di schmittiana memoria che è la persona che sostanzialmente crea, impone lo Stato d'eccezione. Ecco, la magistratura italiana ha imposto al Paese uno Stato d'eccezione e lo ha imposto anche al Parlamento, tant'è vero che il Parlamento contraddice se stesso nel momento in cui rinnega persino quanto

signor Presidente, che in questa Camera i colleghi della sinistra - lo hanno dimenticato - sono minoranza elettorale. Siete minoranza elettorale, 200.000 voti in meno e se non ci fosse stata una legge che vi ha permesso di essere maggioranza, pur essendo minoranza elettorale, ora qui voi sareste minoranza. Per quanto riguarda quella legge, uno dei senatori a vita, che è vostro fiancheggiatore, fu decisivo nell'imporre il collegio regionale

sull'ordine dei lavori, sono costretto a toglierle la parola. Concluda.

è aggiunto" fino alla fine siano sostituite dalle altre: "dopo le parole: "prima fascia" siano aggiunte le altre: ",attualmente in servizio," e che dopo il comma 2 venga aggiunto il seguente periodo: "L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia

Ad integrazione del parere reso sul testo in relazione al comma 11 dell'articolo 3, la Commissione esprime parere non ostativo a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, dell'approvazione dell'emendamento 3.800 (testo 2) come condizionato ai sensi del periodo precedente.»

ai sensi dell'articolo 100 del nostro Regolamento, che esso è frutto dell'elaborazione collegiale della Commissione bilancio. Abbiamo preventivamente preso in esame l'ipotesi che l'emendamento venisse presentato dal relatore e su di esso c'è il parere unanime di nulla osta della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 3.800 (testo 3), come lei ha correttamente indicato, signor Presidente, esso rappresenta rappresenta il contributo della Commissione bilancio a rendere procedibile nel testo quella parte riferita alla possibile assunzione del ruolo di segretario generale della Scuola da parte di un dirigente di prima fascia non appartenente alla magistratura. Se si accoglie l'emendamento 3.800 (testo 3), il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della sul testo approvato dalla Commissione, a proposito della possibilità che un non magistrato sia dirigente della pubblica amministrazione, cade. Sperando di essere stato chiaro, ho terminato.

Presidente, capisco e raccolgo il suo invito alla brevità perché sono state giornate molto impegnative e capisco che i colleghi presenti in Aula vogliano concludere, però

è la riforma di una delle parti fondamentali del sistema istituzionale del nostro Paese e di una delle funzioni più importanti del governo della società inteso complessivamente, cioè

proposti e sottoposti a voto per logiche tutte politiche e corporative dell'una o dell'altra parte: dobbiamo invece ricondurre il senso di questo voto al merito ed ai punti essenziali, e mi limito ad indicarli. Il provvedimento

che molti dai banchi dell'opposizione hanno indicato come uno dei rischi a cui invece noi staremmo esponendo la magistratura con l'approvazione di questo disegno di legge. Io penso che l'aver escluso l'aver escluso la separazione delle carriere e l'aver dato invece un assetto chiaro e rigoroso alla separazione delle funzioni, l'aver eliminato il sistema dei concorsi per le carriere e l'aver indicato invece criteri chiari e definiti per i giudizi di valutazione, l'aver confermato l'autogoverno, l'aver aperto le valutazioni dei consigli distrettuali della giustizia all'obbligo di tener conto dei pareri dei consigli dell'avvocatura, e averle aperte ad altri esponenti laici esterni alla magistratura, siano modifiche che consentono di ricondurre l'ordinamento giudiziario in maggiore coerenza con i princìpi della Costituzione.

interverrò molto rapidamente come i colleghi che mi hanno preceduto. Il nostro voto su questa legge sarà favorevole. È una legge diversa da quella che noi avevamo in mente e diversa da quella che avevamo proposto agli elettori, ma sicuramente è migliore di quella che andiamo a modificare con l'attuale provvedimento legislativo. C'è stato un *iter* abbastanza complesso

le ragioni per le quali il Gruppo dell'Ulivo vota convintamente a favore di questo disegno di legge. Desidero innanzitutto esprimere un ringraziamento al relatore Di Lello, ai colleghi dell'Ulivo che hanno partecipato attivamente ai lavori della Commissione e un ringraziamento particolare al collega Gerardo D'Ambrosio.

l'indipendenza e l'autonomia dell'ordine giudiziario; in secondo luogo; l'efficienza dell'organizzazione giudiziaria; in terzo luogo, la formazione ed il reclutamento, quindi il rapporto tra magistrati ed avvocati. Desidero proporre alla vostra attenzione una considerazione politica che potrà formare ancora base di discussione con i colleghi dell'opposizione

della discussione. La considerazione politica che intendo svolgere è che questa maggioranza e questo Governo conducono in porto una legge così complessa

mentre, con un ben diverso rapporto di forze e con una maggioranza ampia in Parlamento, il centro‑destra nella scorsa legislatura non era riuscito a condurre in porto la sua legge sull'ordinamento giudiziario senza porre ripetutamente la questione di fiducia. inoltre, sottolineare che sullo sfondo delle norme che abbiamo discusso vi è un problema fondamentale per la vita

senza un'organizzazione che garantisca la loro indipendenza e la loro autonomia. Abbiamo lavorato per realizzare questo obiettivo e possiamo, con orgoglio, dire che oggi dal Senato esce un testo di legge ispirato ai princìpi costituzionali e tale da inverarli nella prassi e nell'organizzazione concreta della giustizia. *(Applausi Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, le ragioni di fondo del voto favorevole a questa nuova legge sull'ordinamento giudiziario sono state da me svolte in sede di discussione generale e non ho motivo di modificarle alla luce del dibattito che si è svolto in Aula. Vorrei svolgere tre interlocuzioni: una rivolta al ministro Di Pietro, una al nostro Governo e la terza alla magistratura italiana. Innanzi tutto, vorrei chiedere al ministro Di Pietro, il famoso moralizzatore, di venire presto a rispondere all'interpellanza di cui è primo firmatario il senatore Paolo Brutti, secondo la quale il presidente dell'ANAS da lui nominato, di nome Ciucci, ha una retribuzione complessiva annua lorda di oltre un milione e 500.000 euro, in violazione della norma da noi introdotta nella recente legge finanziaria. Chi ha tutti questi scrupoli di moralizzazione farebbe bene a venire in Parlamento e a rendere conto della propria attività: è vero, non é vero, è giusta una retribuzione di questo genere? Chi è nominato dal ministro di Pietro è esente da ogni forma di controllo di eticità e di legalità? Su questo come su altri aspetti riguardanti la moralizzazione della vita pubblica italiana avremmo piacere di interloquire con il ministro Di Pietro nel momento nel quale, mi auguro il più presto possibile, verrà a rispondere all'interpellanza che è stata presentata.

Ancora una volta in Senato abbiamo risolto un problema difficile, facendo i salti mortali, però vorrei dire, con grande franchezza, che così non va bene. Bisogna registrare la macchina, bisogna dare segnali di discontinuità, bisogna soprattutto che la funzione di indirizzo unitario che la Costituzione e la legge attribuiscono al Presidente del Consiglio si manifesti concretamente e non solo in astratte declamazioni. Io apprezzo il ministro Mastella, pur avendo punti di dissenso con lui da alcuni punti di vista per l'attività da lui svolta: ma un provvedimento di questa rilevanza, la riforma dell'ordinamento di uno degli ordini autonomi dei poteri dello Stato non è solo materia del Ministro della giustizia. Ho visto il Presidente del Consiglio totalmente assente nel momento nel quale un altro Ministro del suo Governo metteva a rischio l'approvazione di questa legge; non ho visto seguita questa legge con l'attenzione che per la sua rilevanza essa merita. E siccome la mia valutazione è che comportamenti di questo genere non riguardano specificamente questo tema, vorrei lanciare un segnale di allarme: attenzione, perché qui non si va avanti a lungo. Non per noi, che faremo il nostro dovere fino in fondo, ma perché in questo modo si logora innanzi tutto un rapporto con il Paese e con i cittadini. La terza considerazione mi permetto di rivolgerla alla magistratura italiana. Non voglio giudicare o esprimere critiche sull'atteggiamento da essa tenuto in questa occasione; mi permetto di interloquire con quella parte dalla magistratura italiana alla quale io, e non solo io, ma tanti di noi, siamo stati idealmente vicini per tanti anni. Devo dire che abbiamo una certa nostalgia di un'Associazione nazionale magistrati nella quale la diversità di punti di vista e di sigle associative esprimeva un effettivo pluralismo culturale, culturale, una battaglia ideale. Essendo io uomo di sinistra, voglio dire che ho nostalgia per Michele Coiro, il giovane pretore di Roma che negli anni del Governo Scelba assolveva la prostituta arrestata per le accuse di oltraggio e resistenza e finiva sotto procedimento disciplinare.

Ho nostalgia di una magistratura che faceva valere i diritti dei cittadini innovando nella giurisprudenza, nel diritto del lavoro, nella tutela del danno biologico*. Ho nostalgia di una magistratura che insieme a noi faceva fronte compatto di fronte alle aggressioni, che ci sono state fino a tempi recentissimi, all'autonomia e all'indipendenza della magistratura ma diceva anche, insieme a noi, che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura non sono il privilegio di un corporazione ma un diritto dei cittadini e, innanzi tutto, dei cittadini più deboli e indifesi, perché se la magistratura non è autonoma e indipendente da qualcuno dipenderà, e non certamente dai lavoratori e dalla povera gente. Mi auguro che anche questa vicenda consenta, all'interno della magistratura associata, il riaprirsi di una discussione su quelle che sono le funzioni ed i compiti democratici, essenziali ed estremamente rilevanti, che si esprimono nella tutela giurisdizionale dei diritti. Mi auguro che si possa davvero voltare pagina.

sono stato definito "autore di un atto vergognoso, irresponsabile e indegno". Sono quindi posto nella condizione di dover chiedere la fiducia

il servizio reso al Parlamento europeo, alla Camera dei deputati e oggi al Senato della Repubblica) ho ancora la dignità di restare qui. Io so che le dimissioni vengono votate a scrutinio segreto. Mi sono informato presso il Segretario generale e mi è stato detto che lo scrutinio segreto è previsto dell'Assemblea. Non capisco bene questo concetto, sarà per il pressapochismo da giornalista, come qualche volta si dice della mia professione di base. In questo caso, essendo stato sfiduciato

Senatore Selva, posso comprendere i contenuti della sua richiesta, ma purtroppo questa decisione non è né nella sua né nella mia disponibilità.